Ricordo agli onorevoli senatori che non abbiano potuto partecipare alle votazioni mediante procedimento elettronico sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del professor Antonio Marzano e di altri coimputati che è possibile dichiarare il proprio voto ai senatori Segretari sul banco della Presidenza.

si pone il problema di considerare se una intercettazione acquisita illegittimamente e che non può essere utilizzata nel processo penale, penale, considerando la diversa natura del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, possa esser utilizzata in sede disciplinare. Il collega Calvi ritiene - e lo ha detto - che la questione sia assolutamente fondata; ha manifestato però una perplessità circa il fatto che la materia possa essere regolamentata nel disegno di legge in oggetto, anziché, più opportunamente, nel disegno di legge già esaminato dall'altro ramo del Parlamento che prevede di disciplinare in modo organico la materia delle intercettazioni.

illegittimamente acquisite non solo non possono essere utilizzate nei procedimenti penali, come già oggi è, ma neanche nei procedimenti disciplinari. Se viene assunto un impegno di questo genere da parte

alla soluzione normativa del problema sollevato. Il relatore, senatore Calvi, ha sottolineato due punti: il primo riguarda i percorsi parlamentari. che interviene su un disegno di legge che il Senato esamina in prima lettura, si propone di modificare una norma che contemporaneamente ci perviene dalla Camera già modificata nel testo sulle intercettazioni,

La seconda considerazione svolta dal senatore Calvi riguarda il contenuto della norma perché, anche se il principio è ineccepibile, il senatore Calvi ha ricordato che i fatti costituenti illecito penale - una soglia di gravità diversa e maggiore rispetto a quella relativa agli illeciti disciplinari. Cosa accade nell'ipotesi in cui da intercettazioni legalmente formulate dovesse risultare che non vi sono gli estremi per l'acquisizione ai fini del procedimento penale e tuttavia risultano fatti che possono essere disciplinarmente rilevanti, fatti cioè che la pubblica amministrazione è giusto conosca per valutare se esercitare o meno la sanzione disciplinare, ma che tuttavia non costituiscono fattispecie di reato? La norma, così com'è formulata, non risolve questo problema. La mia opinione, pertanto, è che, pur riconoscendo la sussistenza del problema, sia per evitare duplicazioni di percorsi normativi sia per approfondire il merito della norma, rispetto alla quale in questo momento per i dubbi che ho dovrei votare contro se fosse posta ai voti, sia opportuna la proposta formulata dal relatore, accolta dal Governo e condivisa testé dal presidente Bianco.

C'è una dichiarazione incondizionata di favore e di fondatezza di un emendamento che riguarda una norma di legge oggi vigente. La circostanza che poi essa sia stata modificata da un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, di cui ancora non è iniziato l'esame nella Commissione giustizia del Senato e che potrebbe anche essere suscettibile

poiché si tratta comunque di intercettazioni che afferiscono ad un processo penale e qui non si intende modificare il disciplinare, è evidente che la tipologia di intercettazioni che possono essere ammesse anche nel procedimento disciplinare non possono che passare al vaglio del giudice, il quale dovrà escludere comunque intercettazioni che attengono alla *privacy* del cittadino e che neppure sotto il profilo disciplinare possono assolutamente essere esaminate. vorrei rappresentare all'Aula la circostanza che comunque, anche in sede di esame da parte del Senato dell'articolo di riferimento che, ancorché modificato dalla legge sulle intercettazioni, nominalmente rimane nel codice di rito, si potrà in questa sede inserire un coordinamento e una modifica del genere. Allora, perché perdere tempo, quando questo disegno di legge entrerà in vigore certamente prima di quello relativo alle intercettazioni, con un lasso di tempo che vedrà tutto ciò che è stato intercettato andare a finire nel procedimento disciplinare con una tutela della *privacy* che evidentemente viene completamente sguarnita delle naturali garanzie?

la circostanza che questo emendamento, oltre alla mia firma, porti la firma di un autorevole esponente della maggioranza. Così come davvero non è di poco conto

in esame è fondato e corrisponde a quelli che sono i principi di civiltà giuridica, si badi bene, non del nostro ordinamento processuale, bensì del nostro ordinamento costituzionale. Ancora, Presidente, procedendo evidentemente

esso riguarda i rapporti tra il processo penale e il processo disciplinare esattamente come nella rubrica del disegno di legge che stiamo discutendo. Con riferimento alla seconda obiezione, vorrei tranquillizzare molti colleghi: il senatore il senatore Calvi ha detto che questo provvedimento tende sostanzialmente a far sì che i soggetti che hanno patteggiato determinate sentenze in sede penale possano essere colpiti sotto il profilo disciplinare. Benissimo. Noi condividiamo perfettamente l'impostazione di questo disegno di legge e faccio presente che l'emendamento in esame non tocca e non riguarda questo punto. Aggiungo che siamo in prima lettura e che, conseguentemente, non vi sarebbe, in ragione di questo emendamento, un appesantimento dell'*iter* parlamentare. La terza ed ultima obiezione del senatore Calvi

in ragione di un disegno di legge che è appena pervenuto dalla Camera. Orbene, per quanto mi riguarda, è chiaro che le leggi si scrivono con riferimento alle leggi in vigore, così così come mi pare sia ugualmente evidente che non si può fermare una legge in attesa che ne entri in vigore un'altra. Vorrei però dire al senatore Calvi: noi, maggioranza e opposizione, siamo perfettamente d'accordo su questo disegno di legge; noi, maggioranza e opposizione, siamo perfettamente d'accordo sulla correttezza di questo emendamento; noi, maggioranza e opposizione, siamo perfettamente d'accordo sulla necessità di intervenire nella specifica materia; non riesco davvero a comprendere la ragione per la quale non lo dobbiamo fare subito, bensì nell'ambito di altro provvedimento, quello che riguarda le intercettazioni telefoniche, che al momento è all'attenzione della 2a Commissione, la cui discussione deve ancora cominciare e in ordine alla quale, per la complessità della materia sono prevedibili emendamenti e correzioni rispetto al testo proveniente dalla Camera. Tutto ciò detto, Presidente, non sono favorevole né a ritirare l'emendamento, né a trasformarlo in un ordine del giorno. Sono dell'idea che, quando si è tutti unanimemente d'accordo nel dire che una determinata formulazione è corretta, questa formulazione deve andare avanti; siccome mi rendo conto che vi possono essere delle necessità di assestamento di pensiero in ordine al punto all'interno della maggioranza, evidentemente - ma questo lo valuterà la maggioranza non sarei in linea di principio contrario ad un eventuale rinvio. Certo è che, per quanto mi riguarda, sono assolutamente contrario sia al ritiro dell'emendamento che alla sua trasformazione in ordine del giorno. Onorevoli colleghi, vorrei brevemente riprendere la questione da quanto, a mio avviso molto correttamente diceva il senatore Salvi, il senatore Salvi, il quale ha fatto una ricostruzione corretta dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista dell'*iter* parlamentare. Siccome non siamo tutti giuristi in quest'Aula, sarà bene ricordare cosa dice l'articolo 268, comma una cosa profondamente corretta ovvero che il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Chi di noi non è favorevole a questa norma e a questo principio? Siamo tutti d'accordo. Il problema che ho posto è di duplice natura. Il primo aspetto - ne converrà, credo, il collega Nitto Palma

Il primo problema riguarda la diversa natura del procedimento disciplinare e del procedimento penale. Tutti conoscono episodi recenti nei quali, in indagini svolte da un magistrato di Potenza, una serie di indagati sono stati prosciolti, ma poi, sulla base di quegli atti, sono stati sanzionati e ritenuti colpevoli dai rispettivi ordini professionali. Cosa significa questo? Che lo strumento e la prova della colpevolezza dell'incolpato e della responsabilità dell'imputato sono totalmente diverse. Si usa quell'intercettazione - penso al problema del calcio per finalizzarla a indagini svolte da organi disciplinari, ma irrilevante potrebbe essere dal punto di vista penale. Ma anche questo è un argomento forse debole. L'argomento sul quale ho accentrato la mia attenzione è un altro. Mi sembra che i colleghi non abbiano riflettuto a sufficienza proprio perché i colleghi della Commissione giustizia, che hanno ricevuto questo disegno di legge, non l'hanno ancora visto o letto. Il problema è il seguente: la Camera dei deputati ha votato pressoché all'unanimità un disegno di legge, che oggi è in Senato alla Commissione giustizia,

Allora, siccome si tratta di un principio importante di garanzia sul quale dobbiamo riflettere e legiferare, la mia proposta quale era? La mia proposta è che l'inserimento in questo provvedimento, che deve essere votato subito perché è urgente votarlo per necessità oggettive, infatti più tollerare che i procedimenti disciplinari possano durare 700 giorni quando 120 giorni sono i termini di prescrizione. Noi dobbiamo approvare immediatamente un provvedimento che è decisivo ai fini di una corretta amministrazione del nostro Paese. questo problema, che pure è importante, risolviamolo subito in Commissione giustizia, affrontando il problema delle intercettazioni e, se vogliamo salvaguardare il principio, approviamo ora un ordine del giorno che dice che questo è un punto importante, che andrà valutato in quella sede, e, nel frattempo, votiamo questo disegno di legge. In conclusione, signor io ho sollecitato un ritiro, che mi sembra ormai sia abbastanza improbabile, ed ho pensato alla formulazione di un ordine del giorno, che non è stato presentato. Si dovrà votare. A me spiace, perché a questo punto ritengo che dal punto di vista legislativo fosse opportuno salvaguardare il principio e, nello stesso tempo, rinviare ad altra norma, che è già presente, la soluzione del tema. Mi sembra che ci sia un'impuntatura, che - devo dire - è pregiudizievole, nei confronti di un principio giusto perché se l'Aula voterà voterà in senso negativo, in qualche modo ci troveremo di fronte ad un voto negativo. Allora, è sbagliato incrinare un principio giusto, ma non è neppure corretto inserirlo in questa norma,

Signor Presidente, mi rendo conto che *ad impossibilia nemo tenetur*. A volte diventa difficile ragionare in quest'Aula, quando si sposano in maniera pregiudiziale delle posizioni rispetto alle quali poi non si capisce come si possa andare avanti. Mi è dispiaciuto molto l'intervento del presidente della Commissione giustizia che, fra le altre cose, ha detto di condividere le affermazioni del collega Guido Calvi, in quanto non era possibile intervenire con un provvedimento che modificava una norma che altro provvedimento aveva già modificato. penale viene soltanto richiamato nell'emendamento in esame e per quanto mi riguarda, signor Presidente, la proposta che le farò alla fine è quella di modificare l'emendamento del collega Nitto Palma (chiaramente con il suo consenso), eliminando tale riferimento. Quello che ci interessa è immaginare che possano essere utilizzati nei procedimenti disciplinari le intercettazioni che sono state in qualche modo convalidate dal giudice e, quindi, che la convalida avvenga così come il codice prevede attualmente; con la procedura del comma 6 dell'articolo 268, con l'acquisizione agli atti o in un altro modo, ci interessa poco. Non è questo il problema.

che è corretto, che, anzi, è un principio di civiltà giuridica che va salvaguardato, ma... Allora, mi soffermo sulle cose che ha detto il collega Guido Calvi. afferma - e questa è una cosa, Guido, che onestamente non mi sento di condividere - che c'è una diversa natura e una diversa gravità tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare.

quando dice che deve esserci un doppio regime perché esiste una situazione più grave, più grave, che comporta l'illecito penale, e quindi il reato, rispetto alla quale devono esserci dei controlli (e per la quale è giusto quindi il controllo del giudice che interviene sull'operato del PM per decidere se si acquisiscano o meno quelle intercettazioni), e una situazione meno grave, che riguarda il procedimento disciplinare. Collega Calvi, lei dimentica che il bene tutelato nell'ordinamento è lo stesso: è il diritto alla riservatezza, è quel diritto a non dover subire un'intrusione violenta che si spiega soltanto - ed è una eccezione - con i presupposti e i requisiti che il codice penale prevede. Quindi, non c'è alcun distinguo tra le due cose e sarebbe assurdo che da una violazione certificata dal giudice del processo penale nascesse un elemento da utilizzare nel procedimento disciplinare. non potrebbe convenire nemmeno il ministro Nicolais, che legittimamente vuole mettere in campo delle scelte che accelerino un percorso che molto spesso è impantanato e non produce effetto: d'altra parte, ogni accelerazione ha dei prezzi

noi stiamo trattando un disegno di legge relativo ai rapporti tra le norme penali e gli effetti sull'azione disciplinare. Ecco perché c'è un emendamento che mette in

c'è un emendamento perfettamente coerente e, se noi vogliamo velocizzare il procedimento disciplinare, ministro Nicolais, dobbiamo farlo rispettando quelle garanzie che sono patrimonio di tutti. Il giustizialismo in questa materia non ci interessa, così come non ci interessa quel garantismo orpelloso - se mi lascia passare il termine - che serve solamente a frenare. Di fronte ad alcuni diritti, però, ci deve essere la capacità, innanzi tutto del Parlamento e dell'Assemblea, di pretenderne il rispetto. Ciò detto, arrivo alla proposta e mi Se il problema è solo formale e nominalistico del richiamo all'articolo 268 del codice di procedura penale (benché non possiamo discutere di un qualcosa che non è una norma, perché c'è stata solo una privazione alla Camera, e quindi non ha diritto proprio

Come verrà regolamentata questa acquisizione è un paradigma astratto che ci convince, nel senso che siamo perfettamente consapevoli che quella regolamentazione, ove venisse modificata e scollegata dai parametri del citato comma 6 dell'articolo 268, sarebbe ugualmente legittimamente applicabile, ma oltre questo mi pare che non si possa andare.

dice:«Ho appena letto il gran bel libro di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo "La casta". Ciò che ora va fatto è tradurre questa eccellente inchiesta giornalistica in misure correttive. E' il nostro vero tesoro nascosto. Si tratta solo di farlo emergere, anche perché non bisogna alimentare un senso di ostilità nei confronti della politica, già troppo diffuso nell'opinione pubblica». Eccellenti parole. Se non fosse che danno l'impressione che il Ministro si sia accorto stamattina del problema. Ho molta stima del ministro Padoa-Schioppa come studioso. Immagino che come tale sia dedito più agli studi che alla lettura delle cronache. Se seguisse le cronache saprebbe che il tema è oggetto di un duro scontro, da qualche tempo a questa parte. Se seguisse gli atti parlamentari, in particolare, saprebbe che è stata presentata, in occasione della legge finanziaria, una serie di emendamenti, a firma mia e di altri colleghi più autorevoli di me, che tendevano appunto a colpire e ridurre per un potenziale ammontare di alcuni miliardi di euro - come dicemmo all'epoca

Mi spiace di parlare di un Ministro che in questo momento non c'è. Ma se per caso e per avventura leggerà gli atti parlamentari, è bene sia reso edotto di questa mia posizione. E vengo alla connessione con il tema di oggi: voterò contro questo articolo perché nell'ultima frase si è aggiunto in Commissione, su iniziativa dei colleghi dell'opposizione e con il consenso del relatore, un periodo per cui si manda una certa documentazione all'Alto Commissario per la prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione. Questa è appunto una di quelle finte autorità delle quali avevo proposto con altri colleghi la soppressione in finanziaria. Per la verità avevo combattuto l'istituzione di questa autorità già nell'altra legislatura. Ho sempre considerato assurdo e persino pericoloso che si volesse combattere la corruzione da un unico centro nazionale, dovendosi contrastare la corruzione e l'illecito con le procure competenti per territorio, con la Corte dei conti competente per territorio, con il controllo politico e sociale nel territorio, con l'iniziativa e la funzione ispettiva dei parlamentari del territorio. Sarebbe un Moloch pericolosissimo quell'organismo

di due vice presidenti, di un dirigente di prima fascia e di alcune unità di personale. Come potrebbe mai questa autorità contrastare la corruzione in tutto il Paese?

Quindi, chiaramente questo emendamento - lo dico in maniera pacata - tende ad occultare l'inutilità di questa struttura, che andrebbe opportunamente soppressa, ed a confortare l'esistenza di una superfetazione istituzionale da eliminare. Ecco perché sono contrario. Non voglio sentirmi dire domani dal ministro Padoa-Schioppa che io, con le mie scelte parlamentari, ho reso più difficile il recupero di quel "tesoro" di cui adesso parla.

e per confutare quanto sostenuto dal relatore. In punto di merito e in punto di sostanza, nel rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, il fatto oggetto del processo penale è lo stesso che Non ci sono fatti circostanti che si aggiungono attraverso le intercettazioni a quel fatto. Si parte dal processo penale, avrà una valutazione penale o sarà ritenuto irrilevante penalmente e sarà valutato in sede disciplinare, ma è comunque una fattispecie limitata a quel fatto. Ecco perché l'irrilevanza che viene dichiarata dal giudice attiene ad una irrilevanza di riferimento al fatto che viene esaminato dal giudice penale e che è identico a quello che verrà esaminato in sede di procedimento disciplinare. Non si tratta, cioè, di circostanze aggiuntive ed ecco perché tutto ciò che è irrilevante attiene a profili di *privacy* che nulla hanno a che vedere con ciò che è oggetto del procedimento disciplinare. in punto di fatto. In punto di procedimento parlamentare, se tutti affermiamo che il principio è giusto e che esso dovrà essere inserito nella legge sulle intercettazioni telefoniche - modificandola, perché non perché non potrà che essere così - allora affermiamo che sappiamo, fin dall'inizio, e ancor più con le modifiche suggerite dal collega Manzione, che evitano il riferimento alla norma, ma che sanciscono un principio di

sosteniamo, in modo assoluto e completo, la modifica sottoposta all'Aula dal collega Nitto Palma.

*(Ulivo)*. Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo voterà in linea con le indicazioni del relatore e del Governo. È evidente, dal dibattito che vi è stato, che questo non esaurirà

D'altro canto, il bicameralismo serve anche a questo e vedere cosa succede nell'altra Camera non è indifferente. La questione esiste, però in questo momento riteniamo che il Governo abbia anche il diritto di vedersi approvato un provvedimento che mette a trasparenza il sistema e che, per certi versi, non ha a che fare con la questione

ci siamo chiesti se la risposta che il Governo voleva dare per rilanciare la pubblica amministrazione potesse iniziare con un provvedimento che è mal visto dalla stessa pubblica amministrazione e dai pubblici dipendenti. Abbiamo ottenuto alcuni chiarimenti da parte del Governo e il nostro voto alla fine, sia pur con qualche perplessità, sarà favorevole. Onorevoli colleghi, i rapporti tra procedura penale e procedimento disciplinare sono collegati in un quadro di princìpi che la dottrina e la giurisprudenza hanno ben precisato.

dovete permettere al senatore Saporito di parlare in un clima meno festoso. SAPORITO *(AN)*. Il secondo principio è che i fatti accertati in sede penale non possono formare oggetto di nuova indagine in sede amministrativa, ma solo sotto il profilo di un apprezzamento diverso disciplinarmente. Il terzo principio è che la condanna dei pubblici dipendenti in sede penale comporta sempre anche il riconoscimento di una responsabilità disciplinare, mentre la sentenza di assoluzione - e questo è un punto delicato - non ha lo stesso valore in sede disciplinare, potendo in ogni caso dar luogo ad una sanzione sul piano disciplinare.

che sposta a favore del procedimento penale l'asse di equilibrio fra azione disciplinare e azione penale, che la giurisprudenza e la dottrina - come avanti ricordavo - hanno chiarito in maniera precisa con dei princìpi che devono dare sistemazione a questa materia.

A mio giudizio, e concludo, signor Presidente, la pubblica amministrazione non ha bisogno di provvedimenti siffatti, ma di un'attenzione maggiore: ci sono i contratti che non si ci sono state le sentenze della Corte costituzionale in materia di *spoils system,* c'è altresì una grande paura e preoccupazione della dirigenza dello Stato; bene, noi non possiamo iniziare soltanto punendo ancora di più, ma con uno sguardo più elevato e con un'attenzione maggiore a quelli che sono i dirigenti dello Stato, ma anche i servitori dell'interesse nazionale.

Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo sul provvedimento in esame perché rende più tempestivo ed efficace il provvedimento disciplinare e risolve una disparità di trattamento tra i condannati con riti speciali e quelli condannati con rito ordinario. *(Applausi

è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 1377, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 1377, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006. Tale Accordo è volto a realizzare un importante atto giuridico di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Congo al fine di favorire investimenti

Tale Accordo è volto a realizzare un importante atto giuridico di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Congo al fine di favorire investimenti già in atto

e al settore delle costruzioni, in quanto è volto a incoraggiare, nel quadro delle maggiori certezze e più precise garanzie che da esso derivano, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle parti contraenti. non esistono investimenti rilevanti effettuati nella Repubblica democratica del Congo da parte di grandi imprese italiane. Gli investimenti esistenti, prevalentemente ad opera di imprenditori italiani residenti nel Paese, sono costretti ovviamente a convivere in condizioni operative estremamente difficoltose. Tuttavia, data la propria rilevanza socio-economica e strategica nel continente africano, dovrà necessariamente rientrare nello spettro delle potenziali destinazioni di investimenti di imprese italiane con proiezione in Africa. Si ricorda che, sul piano politico, il Congo attraversa una fase di transizione in via di completamento, con riferimento alla quale la comunità internazionale nutre fondate aspettative di progressiva stabilità, anche nell'ottica di un progressivo miglioramento delle relazioni con i Paesi confinanti. Nella prospettiva delineata, quindi, l'Accordo in esame è in primo luogo volto a potenziare le relazioni economiche bilaterali e lo sviluppo dell'interscambio con l'Italia, mediante un maggior volume di investimenti, essendo per altro verso destinato ad innescare virtuose dinamiche di sviluppo attraverso il trasferimento di *know-how* tecnologico e manageriale. Nel merito, all'articolo 1, comma 1, l'Accordo definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine investimento. L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo sopra descritto di promozione, stabilisce in capo alle parti l'obbligo di garantire - ritengo molto importante questa parte - un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della Nazione più favorita. All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra parte contraente. L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazione, espropri o misure analoghe. Al riguardo è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Si rileva la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tale organismo nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore. All'articolo 9 dell'Accordo si prevede che le controversie tra le parti contraenti in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un tribunale arbitrale *ad hoc*. All'articolo 11 si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due parti, disponendone altresì, ai sensi dell'articolo 12, l'applicazione anche con riferimento agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore. articoli 14 e 15 dell'Accordo regolano, infine, rispettivamente l'entrata in vigore e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni. Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge. In conclusione, si propone di approvare il disegno di legge e di procedere alla ratifica del documento.

Signor Presidente, lo spirito dell'ordine del giorno G1, che ho presentato insieme al collega Del Roio, riguarda il riconoscimento del fatto che gli investimenti privati esteri possono svolgere un ruolo importante di rilancio e di volano per l'economia di Paesi che che hanno subìto gravi conflitti, come appunto il Congo, reduce da una guerra che lo ha insanguinato per ben sette anni. Un conflitto che però è stato caratterizzato, peraltro, da grandi episodi di corruzione e di sfruttamento illegale di risorse naturali, anche attraverso il sostegno di imprese transnazionali estere. Pensiamo che oggi, attraverso questo Accordo, si possa svolgere un ruolo importante per rafforzare i sistemi di *governance* della Repubblica democratica del Congo, per far sì che

riprendendo e rafforzando gli impegni già assunti dal Parlamento congolese rispetto ai contratti di concessione mineraria e, appunto, alla lotta alla corruzione e agli strumenti di governo dell'economia e dei settori produttivi. Invito quindi il relatore ad esprimere parere favorevole su un ordine del giorno che intende far in modo che questo Accordo costituisca un ulteriore strumento di cooperazione in positivo con quel Paese e con quel popolo.

G1, che contribuisce a fornire un quadro positivo nel quale si colloca questo Accordo. Naturalmente, si tratta di un Paese complesso, che vogliamo accompagnare

l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e *Global Positioning System* (GPS) e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e

che riguardano lo sviluppo dello stesso programma europeo di radionavigazione satellitare ad uso civile Galileo. In particolare, per Galileo si intende il «Programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite», lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all'Agenzia spaziale europea, quale primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. La radionavigazione via satellite è una tecnologia di punta che consente all'utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all'ora esatta, la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine Quanto alle origini del programma Galileo, si ricorda che nel 2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) ha provveduto a costituire l'impresa comune Galileo; dal 2002 al 2005 è stata avviata la fase di sviluppo «2002-2005» seguirà quella di fabbricazione e di lancio di satelliti e l'istallazione di strutture terrestri. Il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo nella sua autonomia presenta due caratteristiche principali: l'apertura a collaborazioni internazionali con Paesi terzi e l'interoperabilità con altri sistemi. In questo quadro, l'accordo con la Repubblica cinese, stipulato nel 2003, si inserisce nella sfera della cooperazione internazionale del Programma Galileo con Paesi terzi.

stipulato nel 2004, è volto ad assicurare l'interoperabilità del sistema statunitense *Global Positioning System*, progettato per scopi militari,

Si ricorda, peraltro, come il Consiglio dei ministri europei dei trasporti abbia enfatizzato nel corso degli anni l'importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di Galileo come sistema globale.

con l'accordo di cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radio-elettromagnetica e il rispetto delle norme relative alla compatibilità per il sistema sicurezza nazionale. Anche per quanto attiene la parte del merito relativa a questo secondo Accordo prego l'Assemblea di prendere eventualmente visione del documento che rassegnerò agli atti della Presidenza. Informo che tutte le Commissioni interessate

Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare come questo provvedimento metta insieme due Accordi, uno con la Cina e l'altro con gli Stati Uniti d'America

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Roberto Petrassi

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Carlo Lancella